Signor Presidente, non è semplicissimo intervenire in mancanza di un quadro definito per ciò che concerne la legge finanziaria, anche se per chi, come me, fa parte della Commissione bilancio, è evidentemente più semplice avere il quadro della situazione. Ad ogni modo, sul bilancio ha detto bene il collega relatore senatore Tecce; condivido soprattutto le sue conclusioni, che ci indicano una prospettiva politica ed istituzionale allo stesso tempo, affinché in futuro la stesura, la lettura e le analisi del bilancio dello Stato siano sottratte a tecnicismi materiali per ancorarsi di nuovo al tema della partecipazione, alla realtà che è sempre e comunque in movimento. Un bilancio dello Stato deve essere qualcosa di più di una relazione ragionieristica, lo può diventare senza perdere nulla in precisione ed esattezza contabile. Della riforma della sessione di bilancio ha parlato diffusamente e con passione il presidente Morando, a cui va anche il nostro ringraziamento per come ha tentato di condurre in porto i lavori della Commissione. Alle sue parole si sono riferiti molti colleghi nella mattinata, tutti hanno condiviso la necessità di un percorso istituzionale che approdi alla riforma della sessione di bilancio che, ridefinendo regole certe, restituisca centralità al Parlamento nella formazione del bilancio, in un rapporto dialettico, non subalterno al Governo. Il nostro Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea concorda su questo obiettivo, con una avvertenza: l'esito negativo del confronto in Commissione trova le sue ragioni più vere nella politica e non nel Regolamento, non ci sono infatti regole che tengano di fronte ad un contrasto politico. Buone regole sono una condizione necessaria ma non sufficiente per raggiungere obiettivi politici condivisi. Oggi in Aula il senatore Morgando non ha potuto svolgere la sua relazione perché questo esito politico-istituzionale non ha trovato concordanza tra le forze politiche, la minoranza può certo giustificare la sua scelta con riferimento alle azioni e alle molteplici iniziative, alcune delle quali all'ultimo minuto, del Governo, anche - lo riconosciamo - con argomenti solidi, ma non può negare che in ultimo la decisione finale è stata sua. La maggioranza ha rispettato le regole, perché è suo dovere garantirne il rispetto, lasciando libera l'opposizione di determinare l'esito finale del confronto. Oggi l'annunciato (o preannunciato) ricorso alla fiducia da parte del Governo, attraverso la voce del presidente Marini, risolve l'*impasse* istituzionale, ma non gli altri problemi. Noi riteniamo che anche il Governo debba riflettere sulla situazione che si è determinata e sulle sue responsabilità, che sono oggettive. Dopo aver innalzato i muri portanti della finanziaria, per utilizzare una metafora cara al Ministro dell'economia, ha lasciato che gli abitanti di questo edificio scegliessero gli arredi in una situazione in cui non è stata chiara la scelta delle priorità. Non si è avuto il coraggio di scegliere priorità condivise, o forse non ce ne erano le condizioni e, in alcuni casi - lo dico con pacatezza, ma con l'augurio che ciò non si ripeta - ci siamo trovati di fronte ad accordi in cui sembrava che al Parlamento si chiedesse una semplice ratifica. Gli esiti del lavoro della Camera, inoltre, ci hanno lasciati molti problemi irrisolti, che con pazienza e tenacia abbiamo affrontato. Se il Governo, come noi auspichiamo e chiediamo, rispetterà i lavori della 5a Commissione e si riferirà anche ai pareri del relatore, che ieri sera comunque ha annunciato proprio nella Commissione che depositerà, per quanto non votato, un documento come riferimento per l'orientamento del Governo sul maxiemendamento,

tutto il disegno di legge della finanziaria, tutta la documentazione e tutti gli emendamenti presentati. Siamo convinti che in quel parere - e, quindi, ci auguriamo nel prossimo maxiemendamento annunciato dal Governo - i cittadini potranno leggere una finanziaria migliorata rispetto a quella licenziata dalla Camera e il Paese potrà riconoscersi in una volontà di dare un'anima - per utilizzare un'altra espressione ricorrente in questi giorni - alla finanza pubblica. Da domani - immagino - potremo entrare nel merito delle singole questioni che qui, questa sera, è un po' difficile anticipare non avendo un testo definito e definitivo a nostra disposizione. Oggi, in effetti, come ho ricordato, il dibattito si è più concentrato sul metodo e sulle regole. Al Governo chiediamo un maggior sforzo unitario nell'individuare i problemi del Paese e nel proporre soluzioni per risolverli. In cinque anni, gli interventi - dico cinque perché noi lavoriamo affinché questa legislatura e questo Governo durino per l'intero arco temporale previsto dalla legge - si possono anche programmare, ma occorre che proponiamo e attuiamo una netta cesura a pratiche che fanno forse parte del nostro carattere nazionale; per cui, alla fine, a prevalere sembrano sempre spinte centrifughe o interessi settoriali. Per noi, per Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, le priorità sono ancora il lavoro, la scuola, la ricerca, la sanità, i diritti e la pace. Con il lavoro come centro della nostra iniziativa politica e la lotta al precariato, in questa finanziaria, nel lavoro in Commissione, abbiamo piantato - uso una metafora - alcuni semi. Abbiamo proposto l'abolizione dei *ticket* sul Pronto Soccorso. Abbiamo proposto un'iniziativa per l'edilizia pubblica residenziale. Abbiamo proposto un rifinanziamento dell'università, una diversa destinazione di alcuni fondi della difesa. Siamo intervenuti sul lavoro. Oggi i giornali fanno riferimento a un'iniziativa unitaria dell'Unione per quanto concerne l'assunzione di altri 200 ispettori del lavoro. Questa iniziativa si basa su un emendamento presentato dal nostro collega, senatore Zuccherini, che appunto proponeva di raddoppiare gli ispettori del lavoro. Questa iniziativa non è settoriale, non è particolare; non solo si richiama all'appello del Presidente della Repubblica affinché questo Parlamento si attivi sul tema delle morti bianche, ma gli ispettori richiamano il tema del lavoro nero, richiamano il tema della relazione tra lavoro e migranti. chiesto, sempre sul tema del lavoro, che per ciò che concerne l'ISTAT ci sia una proroga al 2007 dei contratti di collaborazione e la salvaguardia dei rapporti esistenti. Ci siamo battuti - e speriamo con esiti positivi - affinché sia eliminata la norma che prevedeva l'estinzione delle graduatorie dei precari delle scuole al 2010.

un fondo contro la violenza sessuale e di genere per ciò che concerne il tema dei diritti e l'istituzione di un osservatorio nazionale permanente su questo argomento.

in modo che gli incentivi siano solo ed esclusivamente destinati alle fonti energetiche rinnovabili con conseguente esclusione di quelle non pulite.

Noi guardiamo anche al futuro, più lontano rispetto alla quotidianità. Con l'Unione, lavoreremo affinché questi semi diventino alberi robusti che crescano nel Paese.

alle proteste dei lavoratori che chiedono di riconoscersi in un'azione di Governo che risponda finalmente alle loro esigenze per quanto riguarda la precarietà, il salario, il futuro pensionistico. Abbiamo condiviso le loro ragioni durante la campagna elettorale e riteniamo che abbiano ancora ragione allorché chiedono a questo Governo e alla sua maggioranza di attuare quel programma.

ancor più importanti e significativi di quelli che finora con fatica, ma con una prospettiva futura, siamo riusciti ad inserire nell'attuale legge finanziaria.

onorevoli colleghi, signori del Governo, la discussione svoltasi in Commissione per due settimane è stata approfondita e completa. La maggioranza

le proposte legittime che la maggioranza ha reiteratamente formulato all'opposizione non soltanto sono state rigettate, ma si è verificato che, nonostante l'enorme impegno, non è stato possibile concludere i lavori.

la conclusione dell'esame di provvedimenti complessi e articolati come la legge finanziaria; altrettanto avremmo potuto fare noi negli anni passati. È evidente, infatti, che l'esame

di occultarne la rilevanza; anzi, tutti sottolineiamo la positività di quanto si sta verificando. Tuttavia, la tesi dell'opposizione è che questo incremento notevole, e per certi aspetti anomalo, del gettito,

variazione ai documenti di bilancio per proiettare il maggior gettito sui conti prospettici del 2007 e quindi per incidere

bilancio contenuti nei documenti al nostro esame. Senonché, l'opposizione tace alcuni elementi assolutamente oggettivi che è doveroso reiterare in questa sede e che riguardano sia la destinazione delle maggiori risorse affluite nel bilancio dello Stato nel corso del 2006 sia la problematica della proiezione all'esercizio prossimo venturo delle presunte, in questo caso, maggiori entrate.

ci siamo ritrovati a dover coprire 17 miliardi di euro derivanti dalla nota sentenza sulla detraibilità dell'IVA sulle autovetture. Ci siamo ritrovati inoltre (è uno degli oggetti degli emendamenti del Governo) 13 miliardi di euro di regolazione debitoria per quanto riguarda i fondi delle Ferrovie impegnate negli investimenti, nel corso degli anni, nell'Alta velocità più 17 fa 30), oltre alle *una tantum* che indiscutibilmente sono presenti in questo dato di aumento del gettito (per esempio, quella legata alla rivalutazione delle quote dei cespiti societari, una misura della finanziaria dell'anno scorso), talché tutte queste maggiori entrate sono abbondantemente assorbite da questa pesante eredità debitoria che incide sull'indebitamento fino a sospingerlo al 5,8 per cento del PIL, come è stato anche autorevolmente rilevato in sede europea. È bene che questi elementi siano tenuti nel debito conto perché l'opposizione, ex maggioranza, ha una responsabilità al riguardo. Per quanto riguarda la sentenza IVA, pur provenendo da un dato normativo antico, il Governo italiano, lo Stato italiano, fu diffidato dall'Unione Europea nel 2001 a modificare quella normativa: ebbene, quel Governo, che è stato il vostro Governo, non ha adempiuto, non ha ottemperato per cinque anni, determinando questo peso debitorio ingente. Allo stesso modo, la regolazione debitoria che riguarda le Ferrovie modo, la regolazione debitoria che riguarda le Ferrovie è l'eredità di uno dei tanti strumenti di finanza creativa inventati nel corso degli anni, in base al quale fu attribuita a Infrastrutture SpA, poi fusa con la Cassa depositi e prestiti, una risorsa così ingente non annoverata nei conti dello Stato,

risottolineata questa mattina negli interventi dei colleghi dell'opposizione. Innanzitutto, bisognerà verificare se questo *trend* sarà confermato nel corso del 2007, nel qual caso certamente si determinerà un'influenza positiva sulla finanza pubblica. Ma il Governo ha fatto la stima prudenziale che ha fatto, e bene ha fatto dopo aver conteggiato come dato strutturale i 5 miliardi di maggiori entrate. Ha fatto la scelta che ha fatto perché la differenza, come è noto, non va fatta tra le entrate del 2006

bene. Abbiamo previsto, con la modifica approvata in Commissione all'articolo 1 della finanziaria (una delle tante modifiche migliorative che ci auguriamo il Governo inserirà nel maxiemendamento),

a cosa saranno destinate le maggiori entrate rispetto a quelle previste. Credo che, se il Governo - come ritengo debba fare - accoglierà l'esito della discussione approfondita e rilevante e delle proposte che la maggioranza e la Commissione hanno avanzato in questi giorni, uscirà un testo della finanziaria molto migliore, accettabile e corrispondente agli interessi del Paese.

ai telegiornali ed abbiamo letto le agenzie: ci sono stati autorevoli Presidenti di Gruppi della maggioranza che hanno dichiarato che vi era la necessità di porre la questione di fiducia, perché, da parte dell'opposizione, c'era stato ostruzionismo. Signor Presidente, per carità, è legittimo propagandisticamente dire ciò che si ritiene opportuno fare, però, in quest'Aula, assistiamo quest'oggi all'ostruzionismo da parte della maggioranza ed è assolutamente impensabile che si travisi la realtà in questo modo. Non è un'offesa a noi dell'opposizione; quando riterremo di parlare, parleremo e motiveremo il nostro modo di pensare e il perché dei nostri atteggiamenti. Questa è un'offesa, mi consenta, all'Aula del Senato. A dieci metri da qui si fanno dichiarazioni così pesanti contro l'opposizione e qui dentro si pratica l'ostruzionismo, perché non c'è accordo all'interno della maggioranza sul testo del maxiemendamento da presentare in quest'Aula. Noi abbiamo assistito dal 30 settembre, quando è stata presentata in Consiglio dei ministri la manovra finanziaria, a decine di cambiamenti dei testi, solo da parte della maggioranza, perché non è stato accettato un solo emendamento dell'opposizione; alla Camera prima e in Commissione bilancio del Senato poi, durante i dieci giorni di dibattito. Nonostante questo, il Governo non è nelle condizioni

il Presidente del Senato ad intervenire. Non è consentito che questa mattina i Presidenti dei Gruppi dell'opposizione affrontato - lei era presente, signor Presidente - l'organizzazione dei lavori del Senato con la massima voglia di collaborare (tant'è vero che lo stesso presidente Marini ha ringraziato per il senso di responsabilità dimostrato dall'opposizione) e quest'oggi siamo di fronte a questo scenario. Io chiedo a lei di sospendere la seduta e di chiamare il Presidente del Senato, perché venga qui a riferire che contatti ha con il Governo, a che punto è questo emendamento, cosa ha deciso il Consiglio dei ministri. Riferisca, perché noi non sappiamo se stare in Aula o se uscire, non sappiamo nemmeno cosa dire ai nostri colleghi nel nostro ruolo di Presidenti di Gruppo. Chiedo dunque che si sospenda la seduta, in attesa di conoscere ciò che il Consiglio dei ministri ha deciso questa mattina, se il presidente Marini è in condizione di dirci quando sarà presentato questo maxiemendamento e se siamo in condizione, insomma, di poter regolamentare i nostri lavori, vista la buona

alla luce del fatto che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in Conferenza dei Capigruppo, ha dichiarato che, di qui a breve, il Governo avrebbe posto la fiducia su un nuovo testo di finanziaria.

Avevamo trovato una soluzione che ha dovuto comporre esigenze di rispetto del Regolamento con esigenze di rispetto del percorso che ci eravamo dati. Voglio ricordare come, alla fine, il percorso che ha risolto le nostre obiezioni e ha dato una corretta dinamica ai lavori d'Aula sia stato addirittura individuato dal vice presidente Angius. Ci siamo trovati a lavorare assieme su questa proposta, l'abbiamo modulata, abbiamo individuato una soluzione rispettosa del Regolamento e al tempo stesso rispettosa di questa esigenza.

avviata una discussione generale limitata alle tematiche del bilancio, breve, asciutta, per iniziare, nel pomeriggio, il voto sugli emendamenti e sugli articoli del bilancio e concludere, nella giornata di oggi, questa fase.

non conosciamo. La stessa Commissione, che ha lavorato bene - e colgo l'occasione, l'ho fatto in sede di Capigruppo e lo faccio anche in questa sede, per complimentarmi ed elogiare la responsabilità, la preparazione e la saggezza del presidente Morando, che ha garantito alla Commissione pluralismo di interventi non ha potuto completare i propri lavori sia perché è stata più volte interrotta, nell'ambito della propria attività, da riunioni frequenti che si dovevano tenere tra maggioranza e Governo, sia perché gli emendamenti della stessa maggioranza sono stati ritirati soltanto ventiquattr'ore prima della conclusione dei lavori della Commissione stessa, sia perché non vi erano i presupposti politici per arrivare ad una contemperazione delle esigenze reciproche delle parti, dopo che l'opposizione era stata formalmente invitata dalla maggioranza ad esporre le proprie idee e le proprie controproposte nei giorni pregressi. In ogni caso, la Commissione non ha potuto nemmeno affrontare l'articolo 18, che rimane uno degli articoli preponderanti e più significativi della finanziaria. Quindi, la Commissione, che pure ha ben lavorato,

Devo dire che avevamo ufficialmente e pubblicamente apprezzato non soltanto l'alta mediazione del presidente Marini, ma anche la condivisione delle nostre scelte da parte dei Capigruppo della maggioranza e ci attendevamo, oggi pomeriggio, l'attuazione degli accordi. Mi pare di comprendere, signor Presidente, che così non è, perché assistiamo a interventi continui della maggioranza, che esercita un suo sacrosanto diritto,

come interpretare questo atteggiamento e, conseguentemente, quando arriverà il maxiemendamento sul quale si avvierà la vera discussione generale. Non vi è dubbio, infatti, signor Presidente, che al momento in cui arriverà in Aula il maxiemendamento comporterà innegabilmente lo scivolamento dei tempi della discussione e del voto finale. Questo è conseguente e lo sappiamo, però, in ogni caso, ci saremmo attesi sin da oggi pomeriggio il mantenimento degli impegni assunti in Conferenza dei Capigruppo.

Gli accordi politici si fanno e si rispettano, nella consapevolezza che alcuni vincoli parlamentari non possono essere risolti dagli accordi politici. I vincoli parlamentari si risolvono con modifiche al Regolamento.

È evidente che c'è un problema legato al fatto che il Governo ha preannunciato la questione di fiducia e tuttavia, presso questo ramo del Parlamento, sempre secondo quanto previsto dal nostro Regolamento,

Allora, io credo che dal punto di vista regolamentare la discussione debba e possa procedere così come è stato stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Certo, l'opposizione dice giustamente di non conoscere il nuovo testo della legge finanziaria, ma l'opposizione sa l'opposizione sa - perché in Commissione bilancio una discussione, un confronto penso rigoroso nel merito dei problemi si è svolto - che, al termine dell'esame della Commissione bilancio ieri sera,

Da quel parere evidentemente è possibile avere un'idea di quale sarà il testo che verrà esaminato dal Senato.

Vorrei soltanto aggiungere, in maniera costruttiva, che riteniamo di dover mantenere

procedere ad approvare rapidamente il bilancio per poter dedicare un tempo, degno dell'importanza del provvedimento, al maxiemendamento e quindi ai contenuti della legge finanziaria. Dichiariamo, quindi, che accederemo ad ogni proposta della Presidenza sulla delimitazione dei tempi di discussione

possa interloquire in quella fase, di modo che vi sia una discussione vera sul maxiemendamento che il Governo ha annunziato di presentare. Presidente, noi vogliamo anche rassicurarla, e attraverso di lei vogliamo rassicurare gli autorevoli colleghi intervenuti, che non è nostra intenzione procedere all'infinito nella nostra esposizione di interventi in questa fase. Infatti, il numero degli iscritti

sentito anche il parere del Governo, ci è parso più utile sottoporre all'attenzione della Presidenza una modalità di approccio alle intese raggiunte

vorrei soprattutto rassicurare i colleghi Presidenti di Gruppo che, con molto garbo, hanno posto delle questioni, in merito alle quali, devo dire, in parte hanno anche ragione. Desidero rassicurarli che nella giornata di domani domani daremo il nostro contributo perché si mantenga l'impegno di votare nelle prime ore della mattinata il bilancio e subito dopo svolgere un'articolata discussione sul maxiemendamento, che, nell'interesse del Paese, siamo interessati a svolgere almeno quanto l'opposizione. *(Applausi

Vorrei che non si tenessero più le riunioni dei Capigruppo: se ciò che in esse si stabilisce al mattino non vale più il pomeriggio, significa che sono un rito inutile, una perdita di tempo, e che la disponibilità

e anche dentro le regole; però, io debbo dire che questa mattina noi un impegno politico lo abbiamo preso. L'ho preso anch'io. L'impegno politico è stato, alla fine, di vedere di stringere i tempi per la presentazione del maxiemendamento e di dare assicurazioni all'opposizione, che faceva un'obiezione,

Presidente, la ringrazio. Lei ha ricostruito fedelmente quella che è stata la discussione nella Conferenza dei Capigruppo di questa mattina. però, due aspetti che vanno sottolineati. Il primo - lei non era presente - io ho chiesto di parlare perché nei telegiornali di quest'oggi, i Presidenti dei Gruppi della maggioranza hanno dichiarato che il Governo è costretto a presentare il maxiemendamento e a porre la questione di fiducia per l'ostruzionismo da parte dell'opposizione. Registravamo che l'ostruzionismo lo stava facendo la maggioranza per cercare di perdere tempo, per arrivare a far sì che, *a* *latere* della discussione alla Camera, il Governo trovi un'intesa al proprio interno e scriva questo emendamento.

andava verso la richiesta del voto di fiducia e che il testo presentato e approvato alla Camera non era più da considerarsi definitivo perchè doveva essere modificato. Quindi, abbiamo chiesto, stamani,

Pensavamo che il ministro Chiti andasse in Consiglio dei ministri, si facesse autorizzare a richiedere il voto di fiducia e contemporaneamente portasse il maxiemendamento per poi aprire la discussione.

si parla soltanto per perdere tempo e per dar modo di trovare un accordo all'interno del Governo. A questo punto, quindi, lasciamo l'Aula e torneremo quando ci comunicherete che siete in condizioni di affrontare il dibattito. Ripeto quanto detto nel mio primo intervento: c'è una richiesta, da parte mia, di sospendere i lavori, credo essa debba essere sottoposta al voto dell'Aula, perché c'è un fatto nuovo rispetto a quello che avevamo deciso questa mattina.

il mantenimento di un impegno assunto all'unanimità in Conferenza dei Capigruppo, sotto la sua alta mediazione. Riconosciamo in lei, signor Presidente, il nostro rappresentante anche nelle sue affermazioni e nell'impegno assunto

che apprendiamo essere ancora in fase di elaborazione. Allora, mi chiedo e le chiedo, signor Presidente: visto che il testo è in fase di elaborazione, devo ritenere che il Consiglio dei ministri del Governo Prodi si riunirà nuovamente per autorizzare il Ministro dei rapporti con il Parlamento a porre la questione di fiducia sul maxiemendamento nel rispetto delle procedure a tutela di tutti noi?

continuare a imbastire ulteriori polemiche, perché il dato è oggettivo: non si sta rispettando l'impegno assunto in Conferenza dei Capigruppo. Mi spiace che il collega

Il suo rappresentante in Conferenza dei Capigruppo aveva infatti assunto un impegno. Il collega senatore Ripamonti ci ha ricordato che esistono i Regolamenti e che esistono i diritti dei singoli parlamentari e lungi da noi l'ipotesi di disconoscerli,

da un organismo importante ed autorevole che è proprio la Conferenza dei Capigruppo, che deve essere in grado di guidare i processi formativi delle leggi e le dinamiche dell'attività dell'Aula. dell'Aula. Ho ascoltato con interesse l'intervento - devo dire, più coraggioso - del collega Boccia, il quale ha implicitamente riconosciuto quello che è innegabile, cioè che non si mantiene un impegno, ma che vi è l'impegno, domani (ci auguriamo al più presto), a presentare il maxiemendamento.

mi ha messo un po' in imbarazzo con me stesso l'intervento del collega Ripamonti, al quale riconosco stima ed impegno politico, tuttavia disconoscere così platealmente l'impegno assunto dal proprio Presidente di Gruppo mi fa stare male,

Debbo dire, proprio dinanzi a questo dibattito franco, ma pacato, che noi non avevamo escluso un dibattito,

e credo che, con l'impegno che ho voluto esplicitare e che in queste ore porterò avanti con molta determinazione, possiamo anche andare avanti nel dibattito;

credo che potremmo lavorare positivamente in questo modo e che sia un atto da porre con molta forza dinanzi a chi sta lavorando ora alla definizione del testo, perché di questo si tratta: è chiaro che il Ministro che verrà domani a presentare il maxiemendamento dovrà avere in mano

Questa mattina non è stato escluso che si potesse discutere, nei limiti che sono stati richiamati, ed è stato affermato con forza che il Governo doveva, in tempi congrui, presentare

vorrei dire - e mi rivolgo alla maggioranza in assoluta tranquillità, visto che le cose stanno come ho ricordato - che, se c'è una proposta di sospensione dei nostri lavori e di ripresa degli

Non è uno scandalo accettare di fermarci; vuol dire che da mezzogiorno si inizierà la discussione generale sulla finanziaria, con il più ampio spazio possibile. comprendo benissimo il momento di difficoltà in cui ci troviamo. Credo però bisogna, fra noi, non essere ipocriti. Sono sempre pronto, come i Presidenti di Gruppo dell'opposizione sanno, a riconoscere

per merito anche di un ottimo Presidente della Commissione bilancio, ma anche per merito suo e di tutta l'Aula, è stato costretto a presentare gli emendamenti innovativi rispetto al testo della finanziaria - certo questo crea l'*impasse* - alle ore 20 di giovedì

ha preso atto, ha potuto leggere, studiare e confrontarsi sugli emendamenti del Governo dalle ore 20 di giovedì scorso; dopodiché, il Governo non ha presentato più nulla, checché se ne dica in alcune dichiarazioni fatta all'esterno. Non ha presentato più nulla perché lo abbiamo preteso noi. Si è andati in Commissione bilancio; si è discusso in Commissione bilancio per moltissime ore - come sanno i componenti della 5a Commissione - approvando gli emendamenti